finestra"). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna. **Svolgimento di interrogazioni

In Alto Adige-Südtirol, le associazioni dei commercianti segnalano una frequenza allarmante di questi episodi, con danni economici che arrivano fino al 3 per cento del fatturato. Con la cosiddetta riforma Cartabia, la fattispecie del furto aggravato, da reato procedibile d'ufficio, è stata declassata a reato perseguibile su querela di parte. 625 del codice penale, ha a sua volta l'eccezione delle cose esposte a pubblica fede e cioè la merce in vendita negli esercizi commerciali. Ciò significa che dipende dalla persona danneggiata se la procura e i tribunali sono chiamati a procedere, ma la vittima spesso non è neanche informata del fatto di dover sporgere querela e in tanti casi non è neppure consapevole della differenza tra denuncia e querela. Già prima della riforma i cittadini avevano la convinzione che denunciare non servisse a nulla, posto che la pena detentiva si applica solo per i reati più gravi e che gli autori spesso restano impuniti. A seguito della riforma la situazione è notevolmente peggiorata. In sostanza, anziché rafforzare l'attività investigativa e garantire in modo più rigoroso la certezza della pena, con la riforma si è scelta la strada opposta, vale a dire quella della certezza dell'impunità. Tutto ciò premesso, si chiede di sapere se alla luce dell'evidente incremento del fenomeno su tutto il territorio nazionale, non si ritenga di reintrodurre la procedibilità l'ufficio per il reato di furto aggravato, di cui all'articolo 625 del codice penale,

ringrazio la gentile senatrice. Come sapete, con la cosiddetta legge Cartabia è stato ridotto il numero dei reati procedibili d'ufficio, tra cui quello ed è stato introdotto il principio della preferenza della procedibilità a querela. Ciò per mirare all'effetto deflattivo che dovrebbe ridurre il numero delle pendenze. È stato rimproverato peraltro a questo Governo di averlo in parte vulnerato, cambiando la stessa legge Cartabia fatto un po' di marcia indietro estendendo alcuni reati a procedibili d'ufficio e introducendo nuovi reati. Siamo quindi un po' tra l'incudine e il martello: da un lato, ci si rimprovera di introdurre nuovi reati e di inasprire le pene; dall'altro, invece, come in questo caso, di ridurre quella che è la certezza della pena e la punibilità. Faccio però presente che l'articolo 90-*bis* del codice di procedura penale dà obbligo alla Polizia giudiziaria di informare la parte offesa sulle modalità di presentazione degli atti di denuncia e di querela. Ciò significa che deve anche informare della differenza tra la denuncia e la querela. Faccio anche presente che molto spesso la stessa denuncia, anche se non reca il termine querela, contenendo quella che si chiama la *voluntas puniendi,* è di fatto una querela. In questi casi, quindi, si procede comunque. In ogni caso il Governo avrà cura di accertare nel tempo, anche servendosi degli approfondimenti eseguiti dal comitato tecnico scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sugli altri parametri, e verificare se effettivamente questa riforma, attuata a suo tempo per realizzare quello che di definisce l'effetto deflattivo, abbia avuto un significativo impatto negli aumenti di questo tipo di reati, in modo da poter di nuovo riformare la norma e riportare il reato alla sua originaria formulazione di procedibilità d'ufficio.

capiamo che non è così. Anche se la Polizia e i Carabinieri hanno l'obbligo di spiegare la differenza tra denuncia e querela, sappiamo che le persone pensano, quando chiamano la Polizia, che questa sia già una querela; non capiscono che devono esplicitamente chiedere che venga punito l'autore del reato. Ho visto dichiarare nulle tantissime denunce che non recavano l'esplicita richiesta di punizione.

*(Misto-Az-RE)*. Signor Ministro, in occasione della sua recente visita alla corte d'appello di Brescia per l'inaugurazione dell'anno giudiziario, lei si è dimostrato estremamente attento alla situazione critica delle carceri italiane. D'altronde, il grado di civiltà di un Paese si misura dalla capacità di garantire davvero la rieducazione del condannato, come prevede la nostra Costituzione all'articolo 27. Sono passati undici anni dalla sentenza Torreggiani, con la quale la Corte europea per i diritti dell'uomo ha condannato l'Italia per il trattamento inumano e degradante degli istituti di detenzione. Poco, però, è cambiato e sicuramente non è cambiato in meglio. Noi sappiamo che di problemi strutturali, ma la questione del sovraffollamento - come ella ha giustamente sottolineato - deve essere affrontata. Abbiamo 60.000 detenuti, ma 13.000 persone sono in più rispetto ai posti a disposizione. Questo arreca, ovviamente, un grave disagio alle persone che sono private della libertà, ma è un problema vieppiù grande anche per la Polizia penitenziaria, per coloro che operano all'interno delle carceri italiane. A questa situazione si somma anche la carenza di personale. In particolare, 18.000 sono gli agenti di polizia che mancano all'interno del sistema carcerario. Scarseggiano direttori, educatori, assistenti sociali, magistrati di sorveglianza, personale amministrativo. E questa carenza di personale diffusa ha ricadute pesanti anche sull'organizzazione dell'attività all'interno del carcere, dalla garanzia di regolarità dei colloqui al tema della formazione e del lavoro, che sono così importanti per la rieducazione dei condannati. Vi è poi il bilancio impietoso della sanità penitenziaria, e mi riferisco non solo alla salute fisica, ma anche alla salute mentale. Solo nel mese di gennaio ci sono stati tredici suicidi. Sicuramente la situazione è generale, ma riguarda anche il sistema carcerario bresciano, da Canton Canton Mombello a Verziano. Allora, la domanda è se davvero ci sono quelle risorse, quei 38 milioni, per far fronte ad un ampliamento della struttura di Verziano, e cosa il Governo intenda fare per quanto riguarda Canton Mombello.

il suo intervento e, quindi, anche la risposta. La prima riguarda il sovraffollamento, che dipende ovviamente da due fattori, la capienza carceraria e il numero di detenuti: o aumentiamo il primo o diminuiamo il secondo. Aumentare il primo fattore è molto difficile, perché la costruzione di un nuovo carcere postula un periodo di tempo che è incompatibile con le urgenze. Diminuire il numero dei detenuti spetta, in parte, alla magistratura e anche a un'eventuale ricorso a misure alternative alla detenzione. Però, come vedete anche dalle polemiche odierne, in relazione a un fatto specifico, quando la magistratura, in modo sovrano, applica una pena detentiva, si grida alla incertezza della pena. Noi cerchiamo di intervenire su questo: per esempio, in un primo tempo limitando la carcerazione preventiva. La riforma che all'esame del Senato, devolvendo la competenza della custodia cautelare a un organo collegiale, impedirà quel sistema di porte girevoli che porta alla carcerazione di una persona e alla sua scarcerazione, magari dieci giorni dopo l'arresto, in questo caso aumentando il sovraffollamento carcerario. Per quanto riguarda il suo particolare problema, nell'istituto di pena bresciano verrà realizzato un nuovo padiglione detentivo per 220 posti. L'intervento aumenterà la capienza detentiva dell'istituto senza limitare gli spazi trattamentali. In tal modo si potrà alleviare il sovraffollamento di cui soffre anche l'altra struttura bresciana di Canton Mombello, ormai vetusta e che comunque sarà oggetto di interventi di ristrutturazione. L'intera copertura finanziaria è resa possibile grazie al recente sblocco di 166 milioni di euro, gestiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e destinati a molteplici interventi di edilizia penitenziaria. Segnalo anche che il 6 novembre 2023 si è tenuta presso il Ministero delle infrastrutture la riunione del Comitato paritetico per l'edilizia penitenziaria, proprio sulle attività programmate nell'ambito territoriale di Brescia, al fine di sostenere e superare proprio queste criticità. Per il 2024 è stata assicurata al Prap Lombardia la copertura finanziaria di 2,6 milioni di euro per l'esecuzione del primo intervento, consistente nella ristrutturazione del fabbricato detentivo del braccio destro.

ha messo in evidenza come quella di Canton Mombello sia una delle peggiori carceri a livello nazionale. Quindi, è molto importante che le risorse ci siano e vengano utilizzate. Ovviamente il Comune di Brescia

sicuramente è noto al ministro Nordio, Forza Italia è particolarmente sensibile alla situazione delle carceri italiane, che peraltro è un tema di grande urgenza, tant'è che la maggior parte degli atti di sindacato ispettivo di oggi lo riguardano. Il detenuto è comunque un uomo inerme, la cui salute, sia dell'anima che del corpo, è affidata allo Stato, che credo abbia il solenne dovere di prendersene cura.

del suo mandato ministeriale e ovviamente non poteva essere responsabile del numero *record* di suicidi che si era verificato nel 2022, esattamente 84 suicidi. Nel mio intervento di poche settimane fa, alla sua presenza, quando abbiamo discusso dell'amministrazione della giustizia nel nostro Paese, avevo annotato con grande soddisfazione che i suicidi nel 2023 erano scesi a a 65, quindi un calo molto sensibile rispetto a quelli dell'anno precedente. Quindi, siamo rimasti - io personalmente, ma credo anche lei Ministro, per come la conosco - scioccati dal numero abnorme di suicidi che si è registrato nello scorso mese di gennaio: addirittura tredici in un solo mese, un numero assolutamente enorme, un *trend* che se fosse confermato, ci porterebbe a stabilire nel 2024 un *record* storico assoluto, probabilmente superiore ai 100. Credo che questo non sia nell'interesse e nella volontà di nessuno. Mi pare che anche oggi il presidente

vi siete fatti un'idea sulle cause dell'abnorme aumento di suicidi in questo mese, cioè se c'è un motivo specifico. Non saprei dirlo io in anticipo, ma mi affido alla sua sensibilità e alla sua valutazione. quali iniziative il Ministero e lei personalmente vogliate disporre per cercare di attenuare questo carico così drammatico di eventi suicidari.

un'intollerabile evento al quale bisogna in tutti i modi cercare quantomeno di porre rimedio. Naturalmente, per rimediare a un fenomeno occorre conoscerne le cause. Per quanto riguarda l'aumento allarmante di questo mese, che speriamo venga invece invertito come orientamento nei prossimi, noi non possiamo avere dei dati specifici sulle ragioni di questo particolare momento. Sappiamo però quali sono le cause generali dei suicidi, che sono il sovraffollamento, la tensione e le difficoltà psichiche di alcuni individui. Rispetto a cosa fare,

generale. Prima di tutto, occorre un'azione di coordinamento con le autorità sanitarie locali, con gli enti locali, con le comunità terapeutiche, in modo da individuare, possibilmente sin dal momento dell'ingresso, dell'ingresso, le persone con determinate problematiche che possono condurre a una tendenza suicidaria. In secondo luogo, occorre impartire - e sono state impartite - delle precise indicazioni ai provveditorati regionali e a tutte le direzioni degli istituti penitenziari per creare i presupposti per alleviare in via preventiva le situazioni di disagio delle persone che siano state individuate come soggetti a rischio. Inoltre sono stati stipulati - questa è una novità - dei piani regionali di prevenzione ed è stata implementata l'importante collaborazione con gli ordini degli avvocati, soprattutto con i garanti (ieri abbiamo ricevuto i tre nuovi garanti insediati). È stato anche sottoscritto un protocollo di intesa con il consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi anche questo è importante - per definire un diverso e più strutturato coinvolgimento degli esperti, secondo l'articolo 80, nel trattamento e nell'osservazione di questi soggetti a rischio, e abbiamo anche rafforzato il *budget* per i loro compensi. Sono state fatte delle assunzioni da parte del Ministero nel comparto penitenziario: a titolo esemplificativo, 57 dirigenti hanno già preso servizio e per 224 funzionari giuridico-pedagogici è in corso la perfezione delle graduatorie. Il 26 ottobre 2023 è stato costituito un gruppo di lavoro sugli interventi suicidari ed è emersa la pressante esigenza di rafforzare, anche qui, la formazione del personale. Ripeto, ce la mettiamo tutta per cercare di limitare questo fenomeno che, come già sottolineato, costituisce per tutti noi un fardello di dolore. Naturalmente la prima fase importante sarebbe eliminare il sovraffollamento delle carceri.

soprattutto del Ministro, che conosco da tanti anni, prima in ambito professionale e poi anche in ambito politico, quindi so che le sue convinzioni, come peraltro le mie, sono fortemente ispirate ai valori dell'umanesimo liberale e cristiano. Non possiamo però certamente rassegnarci a questi eventi suicidari come fossero ineluttabili ed imprevedibili, e non possiamo adeguarci a una logica di indifferenza e dello scarto, di cui tante volte ha parlato papa Francesco nel suo magistero. Dobbiamo certamente fare tutti di più ed impegnarci tutti di più. Il problema delle tensioni nelle carceri è assai noto, anche nel carcere di Vicenza che in questi ultimi tempi sta registrando una serie di atti di violenza da parte dei

dovremmo auspicare che queste misure che lei ha indicato oggi siano risolutive e che almeno attenuino un *trend* così drammatico, in modo da non ritrovarci qui fra qualche mese a discutere ancora di un aumento che tutti noi non auspichiamo.

riecheggiano come un presagio sinistro rispetto a quanto all'esterno stava per accadere. Lei aveva parlato di una flessione del numero di suicidi in carcere, rapportando i dati del 2023 a quelli del 2022.

persone affidate alla responsabilità dello Stato si sono tolte la vita. Nel 2022, anno citato dal Ministro quale annus horribilis, i suicidi furono 7, quasi quasi la metà rispetto a quelli attuali. Anche lo stesso Presidente della Repubblica ha sentito l'esigenza di convocare il capo del DAP, il pubblico ministero Giovanni Russo, proprio perché allarmato da questi dati; egli ha espresso in quella occasione la sua preoccupazione. Fa da corollario a tale questione la generale situazione carceraria, laddove, a fronte di 51.179 posti disponibili, vi sono 62.707 reclusi. Il sistema carcerario, quindi, è ancora caratterizzato da un grave sovraffollamento, con strutture e operatori quasi al collasso. Per uscire da questo drammatico *trend* occorrono massicce assunzioni. In legge di bilancio c'era l'occasione di rimediare, purtroppo il Governo si è condannato all'inazione. Il MoVimento 5 Stelle aveva presentato un corposo complesso emendativo, che purtroppo non è stato accolto e che era volto a valorizzare l'esperienza carceraria, al fine dell'adeguamento del trattamento ai canoni della effettiva rieducazione del condannato. Una corposa attività emendativa è stata fatta ultimamente anche con la riforma Nordio. Abbiamo evidenziato l'importanza di alcune figure professionali, come i mediatori culturali e i funzionari giuridici; purtroppo,

proposta in Aula sarà invece accolta. Pertanto, Ministro, si chiede di sapere quali politiche abbia intenzione di intraprendere al fine di offrire adeguata tutela non solo ai soggetti che rivestono posizioni di rilievo all'interno della società civile, ma anche nei confronti dei cosiddetti ultimi, che sembrano scoperti di tutele e quasi dimenticati da questa maggioranza.

dove è stato presentato un programma, assieme a tutta la Rai e a Rai cultura, di distribuzione di moltissimi PC, per portare l'educazione all'interno del carcere, anche dove non è possibile consentire una situazione alternativa a quella dell'espiazione della pena. Abbiamo scoperto oggi che, con questo sistema, 20.000 detenuti su 60.000 hanno iniziato dei percorsi di studio, di formazione professionale

è quello di rilevare la tensione carceraria. Questo avviene ovviamente creando nuovi spazi. Ho già detto che cercheremo di trovarne di nuovi e soprattutto di adattare edifici esistenti e vuoti, come le caserme dismesse. Si sono levate varie critiche: ditemi voi dove possiamo trovare gli spazi nuovi necessari per il lavoro e lo sport, che sono le due attività fondamentali per rilevare la tensione, a monte della quale poi emergono gli episodi suicidari. Dove non ci sono gli spazi per lo sport, per il lavoro e per l'attività fisica all'aperto, può almeno entrare la cultura, può entrare l'educazione, può entrare la vicinanza, che oggi è possibile attraverso la tecnologia e attraverso la telematica, di persone che dall'esterno possono educare. Ci sono 20.000 detenuti su 60.000 che si sono iscritti a questi corsi e che stanno studiando. Stamattina ho visto addirittura delle simulazioni di matematica, davanti alle quali molti di noi esitavano, per per l'importanza e la difficoltà della risoluzione dei problemi posti. È un piccolo, forse un grande passo, verso non dico la risoluzione, ma verso la riduzione di questo drammatico problema, che però transita - lo ripeto per l'ennesima volta attraverso la soluzione del problema fondamentale: il sovraffollamento carcerario. Il sovraffollamento carcerario si può evitare soltanto trovando nuovi spazi che al momento non ci sono, sono, e soprattutto, come stiamo facendo adesso con la nuova riforma, eliminando almeno quelle parti di carcerazione preventiva che poi si rivelano inutili, dannose e dolorose per le persone che vengono incarcerate oggi e magari scarcerate domani.

L'esito, però, in questo caso è diverso, perché noi non siamo soddisfatti della sua risposta. Non tanto perché si possa ritenere che in pochi minuti si riesca ad affrontare un tema così complesso come quello del sovraffollamento o comunque della dignità delle persone in detenzione, ma perché, se sommiamo l'assenza di contenuto della risposta alla relazione che lei pochi giorni fa ha reso in quest'Aula sull'amministrazione della giustizia, ci sembra di capire che ci siano altri interessi dominanti rispetto a quello della tutela dei più deboli nelle carceri, che mirano a tentare di assoggettare il potere giudiziario a quello legislativo ed esecutivo. Sarebbe un disegno lecito,

a seguito della relazione, durante l'intervento del collega Scarpinato, ha deciso di abbandonare l'Aula per non ascoltare quello che si stava dicendo. Comportamento lecito per la maggioranza, per l'opposizione, perché è un modo di esprimere il proprio dissenso. Totalmente inaccettabile e offensivo da parte di chi ha un incarico di Governo; stare seduto su quella seggiola in quest'Aula non è un suo diritto, è un suo dovere. Lei non ha il diritto di stare qui, lei ha il dovere di stare qui ad ascoltare anche quando qualcuno dice qualcosa che non condivide. Peraltro il Regolamento le consente di intervenire in ogni momento nel dibattito. Avrebbe potuto replicare al senatore Scarpinato. Lei non ha offeso il senatore Scarpinato o il mio Gruppo. Lei ha offeso l'Aula del Senato e credo che questo non sia accettabile.

Signor Presidente, signor Ministro, colleghe e colleghi, la legge n. 3 del 2012, la famosa legge salva-suicidi, disciplina una nuova tipologia di concordato per la composizione della crisi da sovraindebitamento di soggetti, persone fisiche e micro e piccole imprese, non assoggettabili alle ordinarie procedure fallimentari. La normativa in vigore disciplina una particolare procedura di composizione della crisi attraverso la quale viene data la possibilità ai debitori che si trovino in perdurante stato di squilibrio economico finanziario, di accedere agli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento, per aderire a un piano di pagamento verso i creditori, al fine di giungere a una soluzione concordata e definitiva della propria posizione debitoria, comporre la crisi ed evitare che essi finiscano nella rete dell'usura e dell'estorsione o, se vi sono già entrati, al fine di aiutarli ad uscirne. Il progressivo rallentamento dell'economia, il conseguente calo dei prestiti bancari alle imprese, secondo quanto emerge da un'indagine condotta dalla CGA, rappresentano infatti i presupposti da cui possono nascere fenomeni di illegalità che coinvolgono in primo luogo le microaziende, spesso a conduzione familiare, che vedono sempre più limitate le loro possibilità di accesso al credito. SOS Impresa stima per il 2023 una crescita del 30 per cento dei casi di usura rispetto agli anni precedenti. Una delle cause di crisi di liquidità delle imprese risiede nella presenza di un apparato burocratico vetusto e farraginoso, non più in grado di rispondere in maniera efficace alle reali necessità delle microimprese e delle famiglie. A ciò si aggiunga lo *shock* economico che ha colpito senza soluzione di continuità il nostro Paese ormai da quasi quattro anni. L'inflazione ha determinato, a parità di acquisti, un incremento della spesa per beni e servizi di 4.185 euro per famiglia, con una conseguente riduzione della propensione al risparmio e un altrettanto conseguente maggior ricorso a prestiti e finanziamenti. In Italia sono sette milioni le persone che si trovano in posizione di sovraindebitamento. un dato rilevante riguarda poi la media dei giorni necessari al compimento della procedura: sono circa 542 i giorni impiegati per ciascuna pratica, ed il 70 per cento di queste non arriva a conclusione definitiva. Il rischio di sovraindebitamento che indistintamente riguarda famiglie e piccoli imprenditori rappresenta oggi una causa di fallimento di molte aziende, già in gravi difficoltà economiche; la gestione delle crisi da sovraindebitamento, soprattutto in una fase economica complicata come quella attuale, si configura, dunque, come strumento avente un'importante funzione economica e sociale, aiutando il consumatore, ed in particolare il piccolo imprenditore, a liberarsi dal peso dei debiti accumulati, a risollevarsi, e a trovare una possibile via d'uscita attività, si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per garantire l'accessibilità alle procedure di sovraindebitamento, rimuovendo gli ostacoli che ad oggi impediscono una più rapida risoluzione delle crisi, per una maggiore tutela della liquidità delle micro imprese e delle famiglie.

Faccio presente, in linea generale, che un Ministro viene addirittura accusato di essere contiguo a formazioni mafiose e quasi di favorire il delitto.

Per quanto riguarda la sua domanda, dal 2015 la direzione generale degli affari interni del dipartimento per gli affari di giustizia, competente alla tenuta del registro degli organismi autorizzati alla composizione delle crisi da sovraindebitamento, si occupa delle attività di iscrizione degli organismi richiedenti, provvedendo a verificare in capo a ciascuno la sussistenza dei necessari requisiti, sia al momento dell'iscrizione sia successivamente, attraverso il controllo sulle variazioni comunicate nel corso del tempo dagli stessi organismi iscritti. Ciascun organismo è inoltre tenuto a istituire un elenco dei gestori della crisi, tra i quali il referente distribuisce equamente gli incarichi, tenuto conto della natura e dell'importanza dell'affare. Il registro in questione conta attualmente 430 organismi scritti, che vantano complessivamente circa 19.000 gestori della crisi. È possibile un'ulteriore implementazione del numero degli organismi autorizzati alla gestione della crisi di sovraindebitamento, sempre che ovviamente gli istanti soddisfino gli imprescindibili requisiti richiesti. Evidenzio anche che la disciplina normativa di riferimento non impone una totale informatizzazione del menzionato registro, perché non sussiste l'obbligo per l'amministrazione di dotarsi di un apparato applicativo informatico di gestione e di definizione delle domande. Pertanto, allo stato attuale, la direzione generale degli affari detiene i dati in modalità cartacea. Su questo aspetto, però, sarà opportuno intervenire perché l'informatizzazione delle procedure certamente può produrre effetti positivi sulla relativa tempistica di definizione. In ogni caso sarà mia cura verificare, per ciò che attiene alle competenze del Ministro della giustizia, l'esistenza di eventuali ulteriori criticità normative che possono incidere negativamente sulla rapida definizione delle procedure. Anticipo sin d'ora, in conclusione, che è in fase di studio presso l'ufficio legislativo un intervento correttivo al codice della crisi di impresa, con il quale si stanno valutando anche alcune modifiche alle procedure di indebitamento volte ad agevolarne l'utilizzo e l'efficienza.

ringrazio per il ricordo, che chiaramente per me è motivo di orgoglio ed emozione. Signor Ministro, la sua risposta ci soddisfa e non avevo dubbi, del resto, è arrivato al successo dopo un fallimento; Bill Gates, prima di inventare Microsoft, ha avuto un fallimento; Elon Musk ha avuto una bancarotta. In Italia, se si parla di sovraindebitati, per non parlare di falliti, si parla di persone morte o vicine alla morte. «Ti amiamo tanto e continueremo a farlo per sempre e a lottare perché nessuno dimentichi che dietro a una persona che ha preso la tua decisione c'era un uomo che poteva essere aiutato».

L'Italia sta vivendo un momento drammatico. Il 17 novembre del 2023 «Il Sole 24 Ore» diceva che 500.000 famiglie hanno la rata del mutuo che è più alta del 50 per cento 400.000 famiglie rischiano di avere la casa all'asta. Bisogna agire subito in due modi: da un punto di vista sociale, di comunicazione, per non far nascere il mostro della vergogna nella pancia di tante persone perbene che non riescono a risolvere il problema dei debiti; in secondo luogo, in punto di diritto, con il codice al quale lei faceva riferimento. Ognuno deve fare la sua parte per evitare che chi va in difficoltà possa pensare a soluzioni come l'usura o il suicidio,

sovranità alimentare Francesco Lollobrigida la questione dei cibi sintetici, su cui questa maggioranza di centrodestra, e lei direttamente, signor Ministro, avete assunto fin dall'inizio della legislatura una posizione molto chiara e netta di assoluta contrarietà. È una battaglia di civiltà per difendere le nostre produzioni di eccellenza, la qualità del cibo che mangiamo, la nostra salute, il nostro ambiente, i nostri agricoltori che - lo ricordo - sono i primi custodi di questa eccellenza. Come ricorderete, infatti, il 17 novembre scorso è stato approvato dal Parlamento il disegno di legge con il quale è stato introdotto il divieto di produzione e commercializzazione di carne sintetica. Lo scorso 23 gennaio 2024 - come è noto - si è svolto il Consiglio agricoltura In quella sede, l'Italia ha presentato un documento formale agli altri Paesi membri, insieme ad Austria e Francia. Con questo documento veniva peraltro richiesto l'avvio di una consultazione pubblica in tutta Europa sulla carne coltivata in laboratorio tutela delle denominazioni dei prodotti alimentari e si chiedeva alla Commissione europea di compiere una valutazione sui cosiddetti cibi sintetici, assumendo una posizione nitida su questo importante argomento. Quando parliamo di cibi sintetici, va sgombrato il campo dagli equivoci. Noi chiediamo che prevalga il principio di precauzione: nessuno ad oggi, infatti, conosce gli effetti e le conseguenze di alimentarsi con prodotti artificiali creati in laboratorio. I dubbi sul cibo coltivato in laboratorio - va detto - sono non solo italiani, ma anche molti altri Paesi. Grazie a questo Governo e a questa maggioranza, che hanno a cuore la tutela della salute dei cittadini e la salvaguardia delle filiere produttive di qualità, l'iniziativa dell'Italia nel Consiglio Agrifish può essere - a mio avviso - uno stimolo verso la definizione di una posizione comune europea su questo importante tema. Considerato che il documento in questione presentato dall'Italia al Consiglio Agrifish è stato anche oggetto di discussione e valutazione da parte dei Paesi membri dell'Unione chiediamo oggi al Ministro di sapere quali siano state le posizioni assunte dagli altri Paesi membri sulla questione del cibo sintetico.

con cui l'Italia è diventata la prima Nazione europea, anzi la prima Nazione al mondo, a proibire la produzione, la commercializzazione e l'importazione di cibo coltivato, sintetico, di *fake food* (in lingua comprensibile al mondo), in difesa del nostro comparto agroalimentare, ma, utilizzando il diritto di precauzione, anche della salute pubblica rispetto ai suoi potenziali rischi. Nel frattempo è stata chiusa la procedura Tris, avviata a seguito della notifica della legge sulla carne coltivata. La chiusura comporta che sia stata definitivamente accertata da parte della Commissione europea la compatibilità della legge con i principi del diritto dell'Unione europea in tema di mercato interno. Diversamente, la Commissione avrebbe proceduto a contestare - come era nelle sue facoltà - le disposizioni a prescindere dalla modalità di notifica. Non ci sarà pertanto nessuna procedura di infrazione né richiesta all'Italia di abrogare la legge. La Commissione chiede solo di essere informata sull'applicazione della legge da parte dei giudici nazionali, con buona pace dei tanti fanfaroni che hanno in queste ore replicato messaggi nefasti, come era avvenuto quando si era sostenuto che questo Parlamento non avrebbe approvato quella legge, che il Presidente della Repubblica non l'avrebbe promulgata, che in Europa saremmo stati isolati. Arrivo quindi all'isolamento europeo. La scelta del Governo italiano è stata oggetto di un documento presentato - come lei ricordava - nel Consiglio Agrifish del 23

e, in particolare, la cosiddetta carne coltivata, rappresentano una potenziale minaccia per l'Europa dal punto di vista sanitario, ambientale, etico, ma anche sociale ed economico. Su 26 Nazioni che potevano sottoscrivere il documento, 14 lo hanno fatto formalmente e altre 5 lo hanno appoggiato in sede dibattito. Il Belgio si è astenuto perché presidente di turno dell'Unione e non è computato ovviamente nel numero dei 26. Si sono aggiunte all'Italia, Austria, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Irlanda, Romania, Slovacchia, Slovenia, Bulgaria, Croazia, Lituania, Lussemburgo, Malta e Cipro. Alcune di queste Nazioni hanno annunciato che presenteranno una legge esattamente uguale uguale a quella che l'Italia ha varato. Siamo però convinti che le nostre posizioni vadano supportate sempre da ulteriori dati scientifici. Non temiamo la trasparenza ed è questa la richiesta che abbiamo fatto all'Europa, di verificare cioè che cosa sta accadendo con operazioni di *greenwashing* che hanno tentato di oscurare i rischi di questo tipo di produzione. Abbiamo altresì chiesto - come lei ricordava - che l'Europa apra rispetto a questi temi

Abbiamo difeso un principio, lo abbiamo fatto insieme. Questo Parlamento ha difeso un prodotto, un modello di civiltà e le altre Nazioni in Europa oggi guardano l'Italia come punto di riferimento in questo senso e ci stanno aiutando a ribadire quei principi che per noi sono naturali. Signor Ministro, mi ritengo molto soddisfatto della sua risposta, innanzitutto perché l'esito del Consiglio Agrifish - come lei ha sottolineato, è stato positivo lo dicono i numeri: su 26 Nazioni, ben 14 hanno appoggiato di fatto la proposta dell'Italia contro i cibi sintetici, che sono potenziale minaccia per l'Europa dal punto di vista sanitario - come citava anche lei - ambientale, oltre che etico, sociale ed economico. Alcune delle 14 Nazioni hanno anche annunciato che presenteranno una legge e prenderanno ad esempio quella italiana approvata da noi in Parlamento. Tutto questo ci dice che l'Italia non solo non è isolata in Europa, ma è prima addirittura, anzi diventa modello per gli altri Paesi. L'Italia è protagonista in Europa, assumendo un ruolo attivo e di primissimo piano nella difesa della qualità dei prodotti dei nostri territori e quindi delle eccellenze agroalimentari italiane. Oggi è grazie all'azione all'azione che lei, signor Ministro, sta facendo, che possiamo portare avanti una battaglia che noi riteniamo giusta anche nel contesto europeo, in un'Europa dove siano i popoli, quindi i cittadini europei, a decidere il proprio futuro e non l'Europa dei burocrati e dei Palazzi.

in principio ci sono state le sue perle di saggezza: la paura della sostituzione etnica, i poveri che mangiano meglio dei ricchi. Poi siamo passati alle azioni, azioni con le quali lei obbligava un treno Frecciarossa a una sosta straordinaria per ragioni personali, comunque non previste dalla normativa e dalla disciplina di riferimento. Poi, lei è tornato al pensiero e ci ha voluto in qualche modo deliziare: per esempio al TG1, quando comunicava al colonnello Villadei, in collegamento dalla stazione spaziale internazionale, il fatto di poter esportare nello spazio, in qualche pianeta futuro, la pastasciutta al sugo e i prodotti tipici italiani. Infine, ma qui non c'è nulla da ridere, l'abbiamo potuta apprezzare quando ha dichiarato di non poter prendere posizione sulle agghiaccianti immagini della nostra concittadina Ilaria Salis, perché non le aveva viste: immagini che ritraevano la nostra concittadina in catene in tribunale. Signor Ministro, mentre lei in qualche modo ci deliziava di questo straordinario contributo politico che ho appena descritto, nei vari mesi del suo mandato, tra una *gaffe* e l'altra, lei ha anche aumentato le tasse agli agricoltori per 250 milioni. E nel mentre che aumentava le tasse agli agricoltori, arricchiva di due milioni il suo *staff* al Ministero. Sarò molto chiara, signor Ministro. Intanto, le chiedo quando inizierà davvero a occuparsi del tema dell'agricoltura in questo Paese. In secondo luogo, se non pensa che sia venuto il tempo di diminuire le tasse agli agricoltori, quegli agricoltori che sono in difficoltà, difficoltà derivanti da problemi molto seri, per esempio la crisi nel mar Rosso, su cui è auspicabile che lei attivi un tavolo. Penso anche al fatto che in questo momento sono in atto forti cambiamenti climatici, che obbligano il settore dell'agricoltura a ripensarsi e chiedono che questo Governo faccia qualcosa per loro e non aumenti le tasse. Attendo la risposta, signor

In sedici mesi di Governo abbiamo dato centralità al settore agricolo in Italia, compiendo scelte che hanno come obiettivo la tutela del reddito e la crescita dei nostri agricoltori e pescatori. Ci saranno più di dieci miliardi per la ripresa degli investimenti, la transizione energetica e la promozione del *made in Italy* e dell'agroalimentare nel mondo, settore cui servono anche le campagne promozionali. Tali campagne ci vedranno protagonisti su tanti giornali ed avrò modo anche di inviarle, avrà la pazienza di leggerle: così vedrà che i nostri prodotti nel mondo sono apprezzati; e più li raccontiamo in ogni sede e più riusciamo a farne capire l'importanza. *(Applausi)*. Abbiamo considerato prioritaria la gestione delle emergenze, sostenendo i settori in crisi, come ad esempio le pere ed i kiwi. Abbiamo scelto di dare priorità a un fondo di 300 milioni per le emergenze, più di quello che corrisponde all'Irpef, ma ci arriveremo. Quello che non potevamo fare in sedici mesi era recuperare totalmente la debolezza in cui questo settore versa per le politiche ideologiche fallimentari messe in campo dall'Unione europea *(Applausi)*, che voi tanto difendete nell'attuale composizione, e che ha erogato su siti sempre più bassi per non coltivare, all'assurdo; che impone regole inattuabili per le imprese, se non con una perdita di produzione tale da non garantire loro la sopravvivenza, costringendoci peraltro a comprare da Paesi terzi che non rispettano i diritti dei lavoratori, dell'ambiente evidentemente ci fanno anche concorrenza sleale. Quando questo è accaduto, voi sostenevate le politiche europee e ciecamente le avete condivise tutte e ancora oggi ammettete di farlo. Oggi le cose sono cambiate: il nostro Governo difende i produttori, difende gli agricoltori e sta dalla loro parte. Un Governo è costretto a scegliere come utilizzare le risorse disponibili e, quindi, sull'esenzione Irpef guardiamo i dati: è un provvedimento per il 60 per cento, interviene in modo orizzontale sugli agricoltori. Quelli che fatturano entro i 50.000 euro ne beneficiano mediamente per 60 euro al mese; l'altro 40 per cento, cioè quelli che hanno un reddito superiore ai 50.000 euro fino a diversi milioni, non la pagavano come gli altri e non si capisce che differenza ci fosse con altri lavoratori italiani che producono, hanno la possibilità di sostenersi, ma pagano l'Irpef. Ne beneficiano dunque più quelli che hanno meno bisogno e meno quelli che hanno bisogno: basta studiare i dati.

presieduto organismi sovracomunali, sapete bene quanto sia importante avere persone assunte nell'apparato pubblico che permettano di efficientare il lavoro di un Ministero. Il MASAF era un Ministero di seconda categoria, purtroppo, e non lo dico per le persone che ne hanno occupato la guida, ad esempio la sua collega Bellanova, che si era resa conto più di voi di quanto fosse importante rafforzare

e le ricordo che il gabinetto per il 72 per cento è formato di impiegati pubblici e noi abbiamo tenuto in grandissima parte quelli che già c'erano prima, perché li abbiamo considerati validi e degni di attenzione e valutazione ulteriore, al pari degli altri Ministeri, che sono stati tutti, anche in termini economici, sostenuti in maniera ben diversa. Basta guardare e compararli. Sono valutazioni. Sono stata anche clemente. Il Governo Renzi aveva stanziato, signor Ministro, 560 milioni, di cui 301 per i coltivatori diretti e 258 per gli imprenditori agricoli. Voi queste risorse le avete tagliate - è la verità, Ministro - causando inevitabilmente, come conseguenza, un aumento delle tasse degli agricoltori. Può girare intorno alle questioni quanto vuole, può leggere tutti i *curricula* di tutti quelli che sono qui, ma questi sono i fatti. Aggiungo, Ministro, che lei farebbe bene a non offendere ulteriormente gli agricoltori, perché lei ha dichiarato che, tutto sommato, non ne avevano bisogno. Io penso che un giro, per rendersi conto della situazione nella quale davvero versano gli agricoltori, sarebbe più che gradito. Non solo, Ministro: lei ha anche lei ha anche non rifinanziato nella legge di bilancio il Programma triennale della pesca. Anche qui sto al merito: stiamo parlando di uno dei settori più fragili, di uno dei settori più fragili, che hanno più bisogno di aiuto e anche in questo caso, piuttosto che rafforzare il suo Ministero, penso che avrebbe potuto avere un occhio di riguardo nei confronti di questa categoria. Mi riservo all'ultimo solo un'osservazione rispetto alle cose che ha detto. È vero: io mi sono occupata tanto di trasporti: ha ragione. Io non l'ho mai visto un Ministro

del nostro territorio. Personalmente, sono figlio di una famiglia di contadini e uso questo termine con orgoglio *(Applausi)* per quello che la terra rappresenta per le nostre donne, per i nostri uomini e per i giovani che oggi si apprestano a questo durissimo mestiere; un lavoro che negli ultimi anni, per una serie di congiunture geopolitiche e di scelte anche operate dal Governo, è diventato sempre più difficile. I costi di produzione sono aumentati ed è sufficiente vedere quanto costava il gasolio agricolo nel 2021 (0,45 euro, mentre oggi costa un euro); quanto costano i concimi; quanto costano i fitofarmaci; quanto costa alle imprese il ricorso al credito che hanno assunto in questi anni per far fronte ai propri investimenti; ciò a fronte di una crescita dei tassi di interesse che supera anche il 50

I prezzi dei cereali sono in crollo vertiginoso e l'ortofrutta è falcidiata dalle gelate e dalle siccità. Cito anche la zootecnia e ricordo che il settore ovicaprino non esiste più, anche a causa delle predazioni: un tema ad oggi non risolto, nonostante siano passati sedici mesi dall'insediamento del Governo. Sappiamo tutti cosa significa oggi tenere in piedi un allevamento, perché gli animali mangiano anche il sabato e la domenica, non conoscono feste, non conoscono estati e inverni. In questo contesto ci sono dei dati e una serie di scelte che anche il Governo ha preso rispetto alla legge di bilancio: quella di non rinnovare l'esenzione Irpef, di cui si è già parlato; l'azzeramento dell'esenzione contributiva per due anni per gli *under* 40; l'imposizione del pagamento dell'assicurazione obbligatoria; la contrazione del credito d'imposta sui carburanti. alcun intervento per accise, costi energetici e delle materie prime. Per tutta una serie di motivi, oggi il reddito delle imprese è a rischio. Troppo poco vengono pagati i prodotti all'origine e troppo costano sugli scaffali. C'è qualcuno che mangia sulla pelle degli agricoltori, delle donne e degli uomini che lavorano e sudano *(Applausi)*, così come delle famiglie che non riescono più a fare la spesa. Per questo motivo, chiediamo quali sono le azioni che il Ministro intende intraprendere per garantire il giusto reddito agli agricoltori con un prezzo equo all'origine ed evitare le speculazioni della filiera. quali sono le azioni che intende intraprendere per garantire maggiore liquidità alle aziende agricole a fronte dell'aumento del costo degli interessi sugli investimenti.

di fare l'opposizione ed io apprezzo il suo modo per la serietà derivante anche dal territorio dal quale proviene e dalla competenze che ha assunto facendo il sindaco di un Comune straordinariamente importante per l'agricoltura. mi permetta però di precisare subito, rispetto alla sua interrogazione, che nella legge di bilancio non è stata introdotta alcuna assicurazione obbligatoria a carico delle imprese agricole. Anzi, al contrario, abbiamo dovuto sanare un buco di 200 milioni riuscendo a garantire con fondi ministeriali il mantenimento in linea con gli anni precedenti del contributo agli agricoltori per la stipulazione delle assicurazioni agricole. Come sa, 200 milioni non è facilissimo trovarli rispetto a un buco causato nel passato, ma lo abbiamo fatto per non far ricadere questo danno sulle aziende già in crisi. Colgo l'occasione per dire però che il sistema assicurativo - così come l'avete tenuto in piedi negli anni di Governo - è sbagliato e non ha raggiunto nessuno degli obiettivi che si era posto - sono dati oggettivi - tant'è vero che con le Regioni e con le associazioni agricole lo stiamo riformando. Coordinandoci con le Regioni e con le associazioni agricole, abbiamo intenzione di utilizzare anche un criterio che metta in condizione gli agricoltori di attivare davvero le difese attive e sottoscrivere contratti di assicurazione, perché il 7 per cento di assicurati sul territorio nazionale è davvero un risultato fallimentare di un sistema. In poco più di un anno di Governo abbiamo avviato

parità di risorse disponibili, abbiamo scelto di coprire il buco di cui ho parlato prima, e abbiamo scelto di istituire un fondo per le emergenze. Come lei sa, quest'anno molta della viticoltura italiana è stata colpita dalla peronospora e su questo dobbiamo intervenire. Per quanto riguarda la pesca, dobbiamo intervenire sull'emergenza del granchio blu, perché si ripeterà.

fondi europei per le emergenze. L'Irpef era un intervento orizzontale, che beneficiava di più i ricchi agricoltori, le persone più abbienti, le grandi aziende e molto meno o quasi per nulla quelli che invece hanno difficoltà.

per i finanziamenti agricoli per 80 milioni; le imprese per giovani e donne per 20 milioni, Generazione Terra li ha portati a 60 milioni; i prestiti e gli interventi cambiari per l'ortofrutta sono stati aumentati e abbiamo garantito ulteriori 20 milioni in bilancio; abbiamo quasi raddoppiato i fondi per il PNRR; abbiamo semplificato le operazioni per arrivare a un agrisolare che produca più energia pulita, senza danneggiare l'agricoltura.

abbiamo mantenuto e intendiamo mantenerlo. Oggi la Francia ci viene dietro con azioni strategiche che sono esattamente quelle che noi abbiamo già cominciato a mettere in campo. Grazie per l'ascolto. Avremo tante altre occasioni per confrontarci sull'interesse comune a valorizzare l'agricoltura italiana, che immagino tutti capiscano quanto sia diventata importante,

sembra quasi abbia raccontato che fa il Ministro da un giorno e mezzo. Vorrei dirle che sta lì da un anno e mezzo. Alcune delle risposte che abbiamo chiesto nella nostra interrogazione dovevate metterle in campo questo Governo e lei. Abbiamo avanzato alcune chiedendo più tutela, esoneri contributivi, il blocco delle assicurazioni sulle calamità, la proroga del credito d'imposta per l'acquisto del carburante agricolo. Niente di tutto questo. Ci aspettavamo un avvio di programma di sostegno per aiutare le imprese agricole e gli agricoltori. Ma niente di tutto questo, fino a questo qualche giorno fa. Solamente ieri questo Parlamento ha approvato il decreto energia. Avevamo pensato di presentare degli emendamenti, ma non ci è stato nemmeno consentito. Alla Camera abbiamo provato a migliorare quel testo, per dare aiuto alle imprese e agli agricoltori, ma vi siete girati dall'altra parte. Allora io mi chiedo: questo Governo e lei, Ministro,

gigantesco: qualcuno si è accorto nel Governo e lei si è accorto di quello che sta avvenendo in Italia? Del grido di dolore degli agricoltori? Di tutto quello che il mondo dell'agricoltura grida e chiede al Governo? E allora, se c'è tutto questo, noi chiediamo che il Governo utilizzi un programma complessivo sull'agricoltura, venga in Aula, discuta con le categorie produttive. Insomma, chiediamo che ci sia un grande piano di aiuto per gli agricoltori. Vede Ministro, io penso che in questo momento viene chiesto che lei faccia in fretta, che il Governo faccia in fretta e si muova, probabilmente, ma lo dico senza retorica, perché l'agricoltura, a differenza di quello che lei può pensare, è un treno che non si può fermare.

Negli ultimi quindici anni, infatti, sono diminuite del 37 per cento le imprese agricole: cinque milioni di persone non fanno più agricoltura, cinque milioni di aziende hanno chiuso i battenti. E perché lo hanno fatto in questi quindici Per una serie di errori strategici e demagogici di un'Europa che ha disincentivato la produzione, pensando che si potesse smettere di produrre per acquistare le materie prime in posti dove costava meno, non importava che fossero garantiti i diritti dei lavoratori o le norme igieniche di qualità; un'Europa che non ha saputo coniugare la sostenibilità ambientale con la sostenibilità economica e sociale. Il *green deal* è oggi sotto gli occhi di tutti. Oggi gli agricoltori protestano contro le follie demagogiche dell'Europa, in cui non solo la sinistra è rimasta impantanata, ma ne è anche stata complice. esponenti del PD parlare della situazione nella quale versa l'agricoltura senza fare i conti con il proprio passato mi sembra alquanto ridicolo e strumentale. Ma va bene, ci sta nella narrazione quotidiana. Abbiamo letto di peggio. C'è stata una PAC che da sostegno al reddito è diventata uno strumento demagogico a sfondo pseudoambientalista. E poi, alla fine, sottolineo la narrazione che è stata utilizzata per far passare gli agricoltori per dei grandi inquinatori. Questo aspetto è forse peggiore delle operazioni economiche messe in atto. *(Applausi)*. Si è pensato che fosse l'agricoltore il grande inquinatore. È arrivato questo Governo, quindici mesi fa. Non aveva la bacchetta magica, ma mai come in questi quindici mesi sono arrivate risorse all'agricoltura, tante, anche dal PNRR, per facilitare le produzioni agricole, per non schiacciare il reddito degli agricoltori sulla filiera. Abbiamo iniziato un lavoro difficile, importante, non l'abbiamo concluso. Abbiamo una legislatura davanti, abbiamo quattro anni. Ma, anche se solo pensassimo di mettere le risorse che abbiamo messo in questo anno nei prossimi quattro anni, altro che piano strategico: si tratterebbe di un vero piano economico economico e strategico, cosa che prima non si era mai vista. Dirsi a favore degli agricoltori oggi che gli agricoltori protestano in piazza, quando si è contribuito in maniera devastante alla loro condizione, potrà essere un motivo di *spot* in TV su Rai 3, oppure per far girare i video, ma non legge in realtà la situazione. Quindi noi chiediamo, Ministro, cosa ha fatto in questi quindici mesi e con quale approccio oggi affrontiamo anche le politiche europee?

continuava a chiedere perché non protestassero contro il Governo. Non è il Governo che causa quello che abbiamo patito negli ultimi anni. E quindi perché protestano in Europa? Che cosa è successo nell'Unione europea

coltivare meno significa mantenere l'ambiente più pulito. No, sono gli agricoltori i primi ambientalisti, sono quelli che l'hanno mantenuta la loro terra perché la amano e perché dà loro un reddito. Questa è la verità che dobbiamo riportare alla luce con operazioni oggettive, guardando anche a un fenomeno che ha dell'illogico: se tu diminuisci le tue produzioni, ma il consumo di quegli alimenti resta invariato, vai a comprare quelle merci in Paesi terzi che non difendono i diritti dei lavoratori, dell'ambiente; il mondo non ha confini

più solide, ma nella maggior parte dei casi per abbandono della terra, desertificazione del territorio, spopolamento di alcune aree importanti. In Europa abbiamo sostenuto queste tesi. Noi siamo dalla parte degli agricoltori: sostenibilità ambientale se c'è il mantenimento della produzione; meno agrofarmaci quando ci sono cure alternative o ci sono piante più forti che possano garantire la loro produzione e il loro reddito. *(Applausi)*. L'uomo è un bioregolatore sulle specie animali: dove sono a rischio di estinzione vanno aiutate, ma quando sono troppe, come gli ungulati e i grandi carnivori, anche su base di dati scientifici c'è la possibilità di diminuirle. I nostri agricoltori - e questo ha dato fastidio a tanti - sono uomini e donne libere, che vivono di lavoro e terra, vogliono fare quello e devono essere messi in condizione di farlo. Non chiedono né sussidi né reddito di cittadinanza e noi siamo con loro.

e l'utilizzo di agrofarmaci; lo abbiamo fatto sui crediti di carbonio e sulla legge che prevede che l'agricoltore sia il custode del territorio. A noi fa enormemente piacere che lei abbia fatto firmare anche altri suoi colleghi e sia stato promotore di un documento che rimetteva l'agricoltore al centro dell'ambiente e non in competizione con con esso. È un lavoro duro e lungo. Se fosse stato facile, sarebbero bastati gli altri. Oggi siamo convinti che questo lavoro lo possiamo fare noi, perché abbiamo un approccio che premia la produzione, che vede gli agricoltori come persone che meritano il nostro sostegno. In Italia solo il 3,6 per cento della popolazione lavorativa è impiegata in agricoltura, ma il valore dell'agricoltura va oltre quei 74 miliardi, va oltre i 580 miliardi dell'agroalimentare. È un valore che racconta la nostra storia, universalmente riconosciuta nel mondo, con la quale possiamo considerare i nostri prodotti come veri ambasciatori.

il 1° febbraio del 2021 Tatmadaw, che è il nome con cui viene conosciuto l'esercito birmano, attuò un colpo di Stato, cancellando il Governo legittimo che era stato eletto nel novembre dell'anno precedente. È esattamente in quell'occasione che Aung San Suu Kyi, che era da poco ridiventata Presidente e *Premier* del Governo del Myanmar, torna in galera, rivivendo una storia che aveva ampiamente travagliato la sua vita.

più di 700.000 sono fuggiti nei Paesi vicini, un milione di rohingya sono invece in Bangladesh. Questo determina il fatto che ci il fatto che ci siano in quel Paese oggi 18,6 milioni di persone che sono in condizione di difficoltà

A tutto questo l'esercito ha risposto uccidendo 30.000 civili in 910 bombardamenti aerei che avvengono sulla popolazione civile, in 1.132 attacchi di artiglieria, attraverso 26.000 arresti tra la popolazione e lo sfollamento obbligato di 1.335 villaggi. Forse non abbiamo presente come è fatto il Myanmar, ma si tratta di un Paese che sta tra la foresta e le città e le zone interne periferiche non solo sono ampiamente travagliate da questioni che riguardano anche il rapporto tra le minoranze, ma sono territori nei quali già non c'era certo la ricchezza. la Giunta ha annunciato la prosecuzione di altri sei mesi di stato d'emergenza. Ci sono state molte condanne, anche del nostro Paese. Ci sono condanne sul lavoro forzato, c'è la minaccia dell'ILO di rinviare la Birmania alla Corte internazionale di giustizia, il Gambia lo ha già fatto. Vorrei però chiedere tramite lei, signor Presidente, al nostro Governo, visto che che l'Italia avrà la Presidenza del G7, di utilizzare quell'occasione anche per ricordarsi che c'è la Birmania, che in Myanmar c'è una reazione, che ci sono forze, a partire dal Governo in esilio nella foresta, che stanno cercando di difendere la popolazione e che credo abbiano bisogno che continuino le sanzioni occidentali e gli interventi affinché non si continui a bombardarli da parte dell'esercito che ha compiuto il colpo di Stato.

n. 615 ormai è un ricordo. Parlerò al singolare, ma in questo momento rappresento tutti i cittadini del Sud Italia, o quantomeno chi serba in cuore gli interessi della nostra terra, l'Italia. Ebbene, dal 2001, con artificio tecnico e con tecnicismi burocratici, si sono create le condizioni per concedere ulteriori forme di autonomia, ulteriore inganno per una terra che già risente dell'assegnazione dei fondi statali in base alla spesa storica. Ma cos'è la spesa storica? Chiariamolo: è un inganno. Spesa storica vuol dire che un territorio, un Comune riceve dallo Stato zero euro per i servizi essenziali, dagli asili ai trasporti, solo perché - udite, udite - l'anno precedente era destinatario di zero risorse. Ma di chi è la colpa? Degli amministratori? Certamente no. La colpa è della cattiva politica dello Stato. Hanno sbagliato in tanti, bisogna essere onesti, basti pensare alle responsabilità gravissime di quella bicamerale guidata da D'Alema e Berlusconi, che riformò il Titolo V della Costituzione e che di fatto spalancò le porte all'autonomia differenziata. Preso atto di ciò, è solo una questione di giustizia e di equità. I meridionali rivendicano i propri diritti calpestati da decenni. Infatti, tra il 2001 e il 2017, come conferma Eurispes, la mancata applicazione della clausola del 34 per cento ha privato il Mezzogiorno di circa 850 miliardi di euro. Questo è un vero e proprio insulto all'articolo 3, comma 1 della Costituzione che recita: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge al secondo comma: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale (...)». Per tale motivo, ho depositato un disegno di legge che reca l'obiettivo di ottenere un risarcimento delle risorse sottratte al Sud Italia. sottratte al Sud Italia. Reputo vergognoso che la concessione di ulteriori forme di autonomia si applichi ad invarianza finanziaria quando sarebbe stato giusto ed equo partire dallo stesso livello economico Nord-Sud, così come disposto dall'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, secondo cui occorre ridurre il divario e i livelli di sviluppo delle varie Regioni.

porto una denuncia gravissima e cioè che l'associazione Cittadinanza attiva aveva chiesto al Comitato tecnico scientifico preposto alla definizione dei LEP di venire di venire a conoscenza delle modalità con cui venivano determinati. Il Dipartimento degli affari regionali ha rigettato invece la richiesta, sostenendo che questi verbali sono da ritenersi tra i documenti che afferiscono alla formazione di atti amministrativi e pertanto non soggetti a trasparenza. Eppure ricordo che la definizione dei LEP rappresenta l'unico strumento per non rendere l'autonomia la pietra tombale delle aree fragili del Paese.

valutare che gli interventi che possono essere svolti in sede di discussione generale (ricordo infatti che da poco abbiamo fatto quattro ore di discussione sull'autonomia differenziata)